Segre e Sisto. Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2,

L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna. In data 9 agosto 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze: «Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» (1222).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

Discussione di ratifiche di accordi internazionali II. Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge: 1. Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie La seduta è tolta